ringrazio tutti gli intervenuti perché mi sembra che il dibattito di oggi sia arrivato al cuore del problema e siano stati sollevati in quest'Aula i temi che più propriamente attengono alla ratifica dell'accordo tra Italia e Libia. Voglio ringraziare soprattutto chi - e cito per tutti il senatore Marcenaro - ha voluto ricordare che, nascosto tra le pieghe di questo Trattato, c'è il tentativo di chiudere una storia molto lunga, quasi cent'anni di storia, dal 1911 ad oggi,

Dicevo, è l'occasione per ricordare questo, anche per evitare qualche incidente di percorso, come quello della senatrice Marinaro, il Governo libico non è attento solo al problema degli anni Venti e Trenta, ma più correttamente, secondo il Governo libico, ai problemi nati nel 1911 e durati praticamente fino ad oggi.

dire, a titolo personale, ma anche a nome del Governo, che attorno a questo accordo vi è una carenza di *pietas*, di attenzione ad alcuni aspetti difficilmente quantificabili, che non si misurano in miliardi di dollari, ma che fanno parte della storia dei rapporti tra l'Italia e la Libia. Voglio citare, ad esempio, un problema che non è in questo Trattato, ma che deve restare all'attenzione del Parlamento: il problema dei cimiteri civili in Libia, che ormai ovviamente sono abbandonati. Nel caso di Tripoli rappresentavano - questo sì! - un insulto alla dignità nazionale, che in qualche modo si è provveduto a correggere; dall'altra parte,

che forse avrebbero bisogno di essere più maturati, anche per capire le ragioni della difficoltà di questo accordo, e probabilmente necessiterebbero di qualche atto simbolico che in qualche modo ricordasse giustamente - come sottolineava il senatore De Eccher - che non tutto quello che è avvenuto nei rapporti Italia-Libia può essere buttato via senza alcun commento critico anche sulle posizioni che la Libia ha via via assunto. Come diceva la senatrice Bonino, siamo di fronte a un grande atto di realismo politico; di fronte a cento anni di storia, di contestazioni, i Governi italiani da 15 anni almeno tentano di affrontare e di portare a soluzione questo problema antico, che oserei chiamare di inimicizia fra l'Italia e la Libia. Il risultato raggiunto è soddisfacente; questo è a giudizio del Parlamento. Ho ascoltato con grande attenzione gli interventi non mi pare che vi siano critiche di fondo sulla struttura dell'accordo.

dal Governo libico e dopo l'esperienza coloniale (a dimostrazione quindi che il problema occupa uno spazio molto più ampio), circa 620 milioni di euro. È un problema questo, senatrice Bonino, che il Governo non pensa di risolvere con uno scambio di lettere; esiste una Commissione mista tra il Governo italiano e il Governo libico, che sta lavorando da tempo. C'è una classificazione dei dei crediti, così come sono stati avanzati dalle imprese italiane; c'è l'accordo su alcuni, il dibattito su altri, la negazione di altri ancora.

In ogni caso, è un argomento su cui molto è stato fatto e gli elementi per arrivare ad un giudizio definitivo sono conosciuti. è un'assunzione di responsabilità, a mio avviso, da parte delle imprese, del Governo italiano e del Governo libico, per giungere ad una soluzione, probabilmente salomonica, per evitare che questo processo duri ancora molti anni nel tempo. C'è un problema che riguarda l'immigrazione clandestina, di cui si è parlato molto e rispetto al quale molti hanno attribuito alla ratifica di questo accordo un significato taumaturgico.

D'altronde, nello stesso accordo - se ne è parlato - sono contenute alcune valutazioni che riguardano i confini a Sud della Libia, su cui si è soffermata anche la senatrice Bonino. è vero che il 50 per cento da noi chiesto all'Unione europea non è stato ancora approvato, ma è anche vero che già nel mese di dicembre in Libia si è riunito un comitato tecnico,

che c'è il problema, sollevato soprattutto dall'Italia dei Valori e dal senatore Pedica, della questione NATO. Vorrei ricordare al Parlamento che all'articolo 4 del Trattato,

e preteso dal Governo italiano per poter accedere all'accordo su questo articolo perchè noi riteniamo - lo ritengono anche i nostri avvocati - che il richiamo al rispetto dei principi della legalità internazionale consenta di salvaguardare gli obblighi

la questione delle aziende, dei cinque miliardi e di come funziona, credo che sia ormai una partita acquisita dal Parlamento. Non ho trovato, in senso lato, opposizioni fortemente critiche su questo ragionamento Non mi pare vi siano altre obiezioni sul tentativo di creare un partenariato bilaterale con la Libia. È un problema, come è stato sottolineato, di

e recepisce le istanze provenienti da diversi Gruppi parlamentari. Anche qui voglio ricordare a tutti coloro che oggi si battono per gli esuli della Libia che il Governo non si era dimenticato di questo aspetto quando ha presentato alle Camere questo disegno di legge.

Il Parlamento ha voluto inserire tale argomento all'interno della presente ratifica

Resto comunque a disposizione, qualora nel dibattito sugli emendamenti dovessero emergere altre questioni. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nella discussione generale e - ripeto - resto a disposizione qualora vi fossero ulteriori chiarimenti da fornire.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, da 3.33 a 3.98, da 3.118 a 3.300, da 3.347 a 3.428, 3.1345, da 3.1434 a 3.1490, da 3.2516 a 3.2566, da 3.3595 a 3.3640, da 3.4670 a 3.4710, da 3.6013 a 3.6237, 3.10000, 4.2 e 4.3. Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 4.100, sulla quale il parere è di semplice contrarietà». Onorevoli colleghi, informo l'Aula che è presente in tribuna una delegazione della Repubblica di Cina (Taiwan), guidata dal presidente del Parlamento Wang Jin-Pyng.

giorno G103, il problema è leggermente più complesso. C'è sostanzialmente da parte del Governo un invito al ritiro; c'è infatti un problema di opportunità, in quanto si fa riferimento al rapporto con la Libia e ricordiamo che stiamo parlando in un momento in cui il Ministro dell'interno si sta incontrando con le autorità libiche. Ci sembrerebbe, quindi, di condizionare un rapporto bilaterale

sono stati già verificati a suo tempo; c'è già stato un incarico dei Governi alla Banca italo-araba UBAE. Un aggiornamento di tale ricognizione verrà fatto nelle sedi opportune e dopo le intese che verranno raggiunte dai Governi. Sostanzialmente - lo dico subito - il criterio è se continuare a discutere il complesso dei 620 milioni di euro o se procedere a forme di liquidazioni separate e per importi predeterminati.

Attendo il parere del senatore Barbolini, che se insisterà nella formulazione che viene qui sottoposta troverà un parere contrario del Governo.

Crediamo che continuare ad inserire delle scadenze - che in questo caso sono semestrali - significhi dimenticare che il Governo su chiamata del Parlamento può venire semestralmente, trimestralmente, mensilmente o annualmente.

prevedono una procedura che passa anche attraverso la costituzione di una commissione bilaterale, che possa fungere da elemento di contributo alla velocizzazione delle intese che poi dovranno materializzarsi nell'ambito del Trattato.

in quello che sembra, alla prima ricostruzione dei fatti, un vero e proprio agguato. Due persone su una moto lo hanno freddato.

invita al ritiro

umani scarsamente presa in considerazione dal Trattato. Proprio in questo senso suggeriamo di integrare la Commissione con i rappresentanti di organizzazioni non governative esperte in materia. essendo la partecipazione dei componenti a titolo gratuito, risulterebbe a costo zero per le finanze pubbliche:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «residenti nel territorio dello Stato» vogliamo inserire le seguenti: «rispondenti a tutti i requisiti indicati dalle seguenti lettere».

di esplicitare l'obbligo del possesso di tutti i requisiti indicati dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 per evitare cui una società o un ente commerciale possieda un solo requisito, scatti in automatico l'addizionale all'imposta sul reddito della società.

Ho apprezzato la disponibilità del Governo ad accogliere gli ordini del giorno a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza; tuttavia esprimono un'intenzione per la soluzione di un problema che ormai data da tantissimo tempo. Questo emendamento propone, invece, di cogliere l'occasione dell'approvazione del Trattato per chiudere definitivamente un lunghissimo contenzioso. Questo Trattato rappresenta un atto in sé positivo, in quanto chiude una fase di incomprensioni e di contenzioso tra il nostro Paese e la Libia;

che legittimamente vantano dei crediti nei confronti del Governo libico, per lavori eseguiti dal 1970 al 2002, e che a tutt'oggi non hanno visto ancora minimamente riconosciute le loro legittime aspettative.

l'avvio a soluzione di questo problema, che poi ovviamente dovrebbe trovare una sede e un canale di attuazione attraverso l'intesa tra la parte libica e quella italiana. Lo Stato italiano non può però rinunciare ad un'iniziativa

che la questione è all'attenzione del Parlamento, senza però trovare una soluzione. L'emendamento spinge in questa direzione e sarebbe cosa buona e utile se il Governo vi assentisse e se il Parlamento lo condividesse e lo approvasse.

Gli emendamenti che la delegazione radicale nel Gruppo del PD ha presentato all'articolo 3 del disegno di legge, che poc'anzi il rappresentante del Governo senatore Mantica ha dichiarato essere una parte anomala rispetto alla ratifica di un trattato internazionale,

se prendiamo in considerazione il fatto che con questa decisione salomonica invece di «dividere il bambino in due» lo si è dato tutto a Gheddafi. Ci si preoccupa

regi e fascisti, di cui non dovremmo comunque portare questo tipo di responsabilità. I cittadini italiani, dunque, hanno subito una serie di torti.

150 milioni di euro in tre rate. Il Governo è riuscito a trovare un meccanismo, per certi versi veramente geniale, di finanziamento delle strutture e infrastrutture che sono al centro di questo accordo che, più che Trattato di amicizia, si potrebbe definire

su delle imprese che hanno caratteristiche particolari - ce ne saranno giusto due o tre, l'ENI per prima, che rispondono alle caratteristiche elencate all'articolo 3 - e non si capisce perché lo stesso meccanismo non possa essere utilizzato per recuperare

Alcuni degli ordini del giorno presentati hanno voluto sollevare questo tipo di anomalia, se così la vogliamo chiamare, e il fatto che sia stato accolto l'ordine del giorno G106, di cui sono firmatario insieme al senatore Barbolini, credo che possa lasciare ben sperare sulla possibilità di riuscire a trovare una corsia preferenziale relativamente al reperimento delle risorse economiche e finanziarie per dare seguito fattivo alle richieste al centro di quelle tre proposte di legge. È stata lasciata nelle mani del Governo libico la possibilità

con la tecnica del negoziato sistematico e quotidiano non si arriva mai alla fine del processo e quindi non si arriva mai a dare finalmente i soldi. se potessimo usare un'espressione abbastanza diffusa nel Maghreb, il Governo italiano ha pagato prima di vedere il cammello. Questo è stato stamani da più parti evidenziato. Abbiamo deciso di dare dei soldi ad un Governo che non ha mantenuto una sola promessa, che non ha dato seguito alla firma di un solo patto internazionale, di una convenzione internazionale,

chiedendo di aumentare l'addizionale IRES per recuperare, se non altro, un minimo dei danni che vengono causati da questo Trattato in generale e ridistribuire il danaro italiano a degli italiani. Si è detto, all'inizio della replica del Governo, che si tenta di chiudere un contenzioso avviato nel 1911. Ripeto, siccome non depone a favore della controparte il mantenimento della parola data, se non altro si potrebbe - e abbiamo ancora

per portare avanti questi tipo di iniziative: speriamo che quei soldi non siano stati utilizzati da Gheddafi per comprarsi la Presidenza dell'Unione Africana. Quindi, noi riteniamo che il danno sia già stato fatto e che esistano, purtroppo, non soltanto i numeri della maggioranza ma autorevoli esponenti dell'opposizione principale del Partito Democratico che si sono espressi a favore della ratifica di questo documento, per cui penso che sia pressoché impossibile non arrivare alla ratifica oggi. Abbiamo ritenuto, comunque, di sollevare tutta una serie di questioni per tentare di ridurre questo danno, e l'unico che si poteva ridurre non era certo quello nei confronti dei cittadini libici. A chi parla parla delle malefatte del regime italiano negli anni '10 e del regime fascista negli anni '20 e '30 in Libia, ricordo che sarebbe interessante sapere cosa faccia oggi il Governo di Gheddafi nei confronti dei suoi cittadini: la Libia ha ratificato tutte le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e non ha rispettato una singola virgola di questi documenti. Grazie al fatto di aver sollevato tutte queste questioni alla Camera si è compiuto un passo avanti; chiediamo di farne un altro, recuperando il denaro necessario attraverso questi emendamenti, per poter restituire il mal tolto - credo sia proprio l'espressione adatta a questo tipo di contesto - nei confronti degli esuli e delle imprese italiane scacciati da Gheddafi.

vorrei ricordare che il problema è molto semplice, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo accolto l'ordine del giorno G106 perché ne abbiamo colto lo spirito e la *ratio*, ma non possiamo accogliere l'emendamento. La garanzia sovrana viene data nella certezza che i crediti siano tutti veri ed esigibili,

È ovvio che la terza parte del complesso dei 620 milioni, che è un po' meno della metà del tutto, non vuole disgiungersi dalle prime due parti, per ovvii ed evidenti motivi, poiché ne uscirebbe una sua intrinseca debolezza, cosa che peraltro più volte è stata proposta al Governo italiano. Comprendiamo la *ratio* di questi creditori, che abbiamo più volte invitato a dare anche un termine di fornitura della documentazione. Non credo e non voglio dire qui che il Governo libico si attenga alle regole dell'etica internazionale nella documentazione, questo no; però, sono anni che questa vicenda va avanti. Allora, daremo la garanzia sovrana una volta che saranno accertate le documentazioni e quindi daremo una garanzia di fronte alla certezza che i crediti in discussione sono nel loro complesso tutti esigibili.

E poi ci fermiamo qui, perché è meglio per il Parlamento, per il Governo, per il popolo italiano e per i creditori che esigono questi crediti.

Avverto i colleghi che, qualora venisse approvata la prima parte, potrà essere messa in votazione la seconda parte solo se richiesto da 15 senatori, poiché la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81

Proprio perché è suonata una campana, speriamo che inizi uno scampanio e che, da ora a quando entrerà in vigore questo Trattato,

anche alcuni colleghi del centrodestra, i quali dicono la stessa cosa: bisogna riflettere su quello che è accaduto negli anni passati. Credo che, come ha dichiarato la senatrice Bonino,

in dissenso dal Gruppo, anch'io prendo la parola per ricordare con chi è che noi stiamo facendo un accordo.

vertici dei servizi segreti. L'ex direttore del SISDE, il prefetto Mario Mori, nel 2005, durante un'audizione del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, dichiarava che in Libia i clandestini venivano accalappiati come cani, messi su furgoncini *pick‑up* e liberati in centri di accoglienza dove i sorveglianti per entrare dovevano mettere i fazzoletti sulla bocca per gli odori nauseabondi. Mori parlava di un centro di accoglienza finanziato dagli italiani in Libia, nella località di Seba al confine con il deserto, uno di quei centri di detenzione dove venivano trasferiti anche i clandestini respinti dai centri di permanenza temporanea italiani. Il centro, dichiarava sempre Mori, prevede di ospitare 100 persone, ma ce ne sono 650, una ammassata sull'altra, senza il rispetto di alcuna norma igienica e in condizione terribili. Mori aveva effettuato una visita nel centro di Seba intorno a metà gennaio 2005, cinque giorni prima dell'incontro dell'allora ministro Giuseppe Pisanu con il colonnello Gheddafi;

Tale monitoraggio è finalizzato anche all'adozione di eventuali interventi utili al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. la mancanza di dati certi che indichino il valore esatto dei maggiori introiti derivanti dall'addizionale all'imposta sul reddito delle società, la cosiddetta ENI-*tax*,

e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 al fine di verificare l'effettiva operatività delle misure in esso contenute anche in relazione al gettito atteso dall'introduzione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società. In relazione agli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 30 aprile 2010,

Italia dei Valori, che anch'io ho sottoscritto, pone un altro tipo di problema. Mettiamo che un domani si dovessero esaurire le fonti di gettito per quelle due o tre imprese che sono state classificate come quelle dalle quali vanno prelevati i quattrini con questa addizionale IRES. Cosa succede? Da dove si prendono i soldi per finanziare le grandi opere infrastrutturali? Non si sa. Si è riusciti ancora una volta a dare un lascito: questa è una donazione a fondo perduto da una parte, ma dall'altra non si conosce neanche il fondo da cui si vanno a prendere dei soldi. Quindi, rigettando l'emendamento in esame, il Governo probabilmente ci spiegherà cosa intende invece mettere in atto

al riconoscimento di ulteriori indennizzi in favore di soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti a misure limitative

questi emendamenti possano aiutare il Governo a riparare il torto fatto *in* *primis* da Gheddafi ai nostri concittadini e, in seconda battuta, con la firma di questo Trattato che è riuscito a codificare qualcosa che non era mai stato

italiani, enti e società operanti in Libia e colpiti da provvedimenti adottati dalle autorità libiche. Al comma 1 si prevede la concessione di un ulteriore indennizzo, relativo agli anni 2009-2011,

che con la confisca del 1970 hanno perso immobili, aziende, depositi bancari e pensioni. Da loro abbiamo appreso che la stima minima di un indennizzo decoroso è pari ad almeno 100 milioni di euro. Per innalzare, dunque, lo stanziamento

proponiamo di modificare la copertura finanziaria con riferimento ai fondi - per la verità, esigui - che sono destinati

È chiaro che questa addizionale sarà caricata come sovrapprezzo sulle tariffe che i cittadini italiani saranno chiamati a pagare. del presente Trattato, che dovrebbe garantire la sicurezza delle nostre frontiere e che prevede un impegno finanziario per il nostro Paese di 5 miliardi di dollari

di riconoscimento di ciò che essi hanno subito, potrebbero essere ristorati attraverso il Fondo per interventi strutturali di politica economica,

che chiede soltanto di raddoppiare l'arco temporale entro il quale si possono presentare le legittime richieste di risarcimento. Veramente non si riesce a capire. Mi sembrava di aver colto un moto verso il microfono del sottosegretario Mantica in riferimento a quanto detto prima relativamente ad altri emendamenti. Noto purtroppo che, invece, é stato bloccato. Mi dispiace perché in effetti sarebbe interessante sapere sia per i cittadini italiani che per quelli di altri Paesi ex-colonizzati

della legge 22 dicembre 2008, n.203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.*

ai soggetti titolari di beni e diritti, oltre ad interessi, sottoposti in Libia a misure limitative. Questa è la cifra suggeritaci suggeritaci direttamente dall'Associazione italiana rimpatriati dalla Libia, i quali - come ho detto poc'anzi sempre sostenendo l'emendamento del collega Perduca - hanno perso con la confisca del 1970 tutti i beni in Libia. La stima minima di un indennizzo decoroso dovrebbe essere almeno il doppio di quella indicata:

in un anno si sono visti azzerare totalmente la loro dignità, la loro vita e la loro professionalità. Si sono visti cacciati da un Paese che da amico è diventato nemico nel giro di pochi giorni. Su questo va fatta una riflessione.

stare tranquilli. Con una persona che da trent'anni a questa parte governa facendo il bello e il cattivo tempo - lo abbiamo visto anche con il ricatto dei barconi (perché di questo parliamo)

è un emendamento che deve far riflettere. Verrà da noi condiviso ed approvato ed invitiamo a riflettere anche gli amici del centrodestra: nel

visto e considerato che è stato respinto l'emendamento precedente teso a rendere meno diabolico

un aspetto. Il Governo in questa vicenda - mi riferisco sempre ai crediti - non può avere un atteggiamento notarile. Mi dirà che non ce l'ha; io insisto che non può averlo. Non può semplicemente limitarsi a registrare il fatto che le parti non si mettono d'accordo.

un punto di riferimento per l'applicazione del diritto internazionale. Quindi, sicuramente un qualche problema, anche di carte o di aspetti formali e quant'altro esiste. Occorre un'azione un'azione che aiuti a surrogare le deficienze e le carenze; la richiesta della garanzia di copertura dello Stato sovrano non è una apertura di credito indefinita ma semplicemente una condizione per creare per creare le premesse affinché si possa avere un confronto di merito con la controparte libica, utile a tutelare le imprese italiane. Nessuno chiede che si paghi quello che non si è legittimati a pretendere. Ma è anche vero che forse va fatto uno sforzo comune e che probabilmente lo Stato italiano deve accompagnare le sue imprese in questo lavoro difficoltoso.

È stato detto di no alla possibilità di aumentare la dotazione economica per fare fronte alle richieste legittime di decine di migliaia di italiani, sia che fossero esuli sia che fossero imprenditori, ed è stato detto di no a tre distinte possibilità di recupero del denaro necessario - altri 150 milioni di euro - per fare fronte a tutte queste richieste. Mi pare il minimo che si rigetti quanto contenuto nell'articolo 4 proprio perché, se è vero che è stata inclusa - e so per certo, perché abbiamo avuto più volte la possibilità di

in vigore domani - una anomalia si poteva in qualche modo tentare di mandare un messaggio chiaro ai cittadini italiani e non esclusivamente ad un despota quale Gheddafi è.

non tutti hanno avuto tempo e modo di approfondire la questione: tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, realizzeranno i progetti infrastrutturali di base ovvero importanti opere infrastrutturali, progetti industriali ed investimenti, dovranno essere individuate in ossequio alla normativa comunitaria vigente in Italia in materia di scelta dei contraenti». Mi pare il minimo che si possa previsione all'interno di un testo che ha escluso qualsiasi tipo di buon senso codificato in diritto nazionale ed internazionale, tolta quella frase ad effetto della legalità internazionale. bisognerà che le imprese italiane che andranno a costruire infrastrutture in Libia siano selezionate attraverso una gara di appalto. Mi pare il minimo, visto che poi i terreni dove andranno a edificare potranno essere in qualche modo espropriati con modi e utilizzo, forse, chissà, di denaro anche italiano da parte del regime libico che a noi non sarà possibile controllare perché abbiamo deciso che il Parlamento e comunque anche l'opinione pubblica, visto il silenzio mediatico che è stato dedicato a questo tipo di ratifica,

appalto. Ancora non abbiamo saputo quale sia l'orientamento del Governo sulla questione; speriamo che anche in questa fase possa avere un sussulto di attenzione alla legalità nazionale piuttosto che a quella internazionale, visto e considerato come l'hanno codificato all'interno del Trattato.

come avverrà l'assegnazione e l'individuazione dei soggetti che realizzeranno le opere. Se nel trattato si dice che verranno affidate ad imprese italiane - e la cosa è di grande interesse: la la consideriamo come una boccata di ossigeno per le aziende italiane - chiediamo di valutare quale sia la modalità di assegnazione, anche perché l'applicazione del diritto italiano ci imporrebbe la gara europea.

Torniamo ancora una volta a parlare di copertura finanziaria: ne abbiamo parlato a lungo in questo pomeriggio,

capisce perché, tra tutte le date possibili, sia stato scelto il 30 agosto per firmare questo documento. Il Parlamento non era in sessione, quindi anche volendo non ci sarebbe stata la possibilità di affrontare la questione. avere sotto gli occhi la bozza di ciò che si stava per portare alla firma di Gheddafi, probabilmente si sarebbe riusciti a limitare ulteriormente i danni. Voglio anche far notare che l'ultimo articolo del trattato istituisce il

sull'articolo 6, purtroppo, devo esprimere un voto in dissenso dal Gruppo del Partito Democratico. L'articolo 6 è quello che stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.* Avendo presentato in fase di dibattito in Commissione oltre 6.000 emendamenti ed essendo riuscito a portarne almeno una trentina in dibattito in Aula, è chiaro che il mio voto è contrario anche su quest'ultimo articolo. Starà al buon cuore di tutti i presenti in Aula, oltre che commentare a microfoni spenti ciò che si dice, anche passarsi una mano non dico sulla coscienza - che è una questione che con la politica viene spesso tirata in ballo a sproposito sul proprio manuale di diritto internazionale, se lo hanno, perché con la ratifica di questo documento si è strappata una buona metà di quello che era conosciuto come diritto internazionale,

«Non sono rapporti personali, sia chiaro, ma tra Stati e Governo, i rapporti che non impediscono all'Italia di esprimere le sue posizioni di dissenso rispetto alle decisioni della Russia». Questo vuol dire che bisogna allargare la decisione al

Signora Presidente, colleghi, attendo

Preannuncio il voto favorevole dei miei colleghi del Gruppo Misto e, in modo particolare, della componente dell'MPA, perché riteniamo che quest'accordo si inserisca in modo coerente con il contenuto ed i principi della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e aggressione: in questa scelta della nostra Carta costituzionale vi è anche un giudizio esplicito sul nostro passato.

segnata da lutti e repressioni che hanno giustificato il risentimento di quelle popolazioni nei confronti di quel fatto storico. quindi, che con quest'accordo si ponga fine a quella vicenda e si esprima un giudizio di piena assunzione di responsabilità, con quel principio di continuità che deve caratterizzare gli Stati al di là dei regimi politici che li governano.

con lo Stato libico per fronteggiare insieme il drammatico fenomeno dell'immigrazione clandestina. Ambedue le ragioni, quindi, a mio avviso, legittimano l'approvazione del provvedimento, però vorrei sviluppare un'ulteriore riflessione. Questo potrebbe essere, per così dire, un passo ancora più coraggioso da parte del nostro Paese per costruire una politica di cooperazione, pace e sviluppo che abbia nel bacino del Mediterraneo il centro nevralgico dell'interesse nazionale. Amici del Governo, noi siamo inseriti tra i Paesi fondatori dell'Unione europea, che ha conosciuto un allargamento straordinario e che ha scelto come sua direttrice di sviluppo in modo particolare l'Est l'Est per suturare una ferita drammatica qual è stata la cortina di ferro, ma anche per ragioni economiche e civili della storia del continente europeo. Oggi l'Europa deve volgere lo sguardo a Sud, Sud, perché ha l'interesse strategico di considerare il Mediterraneo un'area di intervento primario e in questa scelta, che ha la ragione fondamentale in una politica di pace, per disinnescare micce pericolosissime di intolleranza religiosa, che trovano la propria ragione essenziale anche in condizioni economiche di fortissimo ritardo nello sviluppo del continente africano. La frontiera dei Paesi del Nord Africa è strategica e l'Italia può rintracciare davvero un fortissimo interesse nazionale se riesce ad imprimere alla politica dell'Unione questa direttrice, di partenariato euromediterraneo di Barcellona, con l'avvicinarsi dell'area di libero scambio, non siano un'occasione retorica, non siano alla fine un'occasione perduta. Lo dico quale persona che crede a una funzione specifica della politica estera italiana e dentro questa funzione particolare anche ad una ragione essenziale per il Sud del Paese. se questo accordo avrà valore, se si confermerà nei suoi contenuti attraverso lo sviluppo di queste relazioni privilegiate (che hanno anche delle controindicazioni, perché interferiscono in qualche modo anche con

l'impegno del nostro Paese a sviluppare questa politica di cooperazione e di sviluppo che abbia verso il Nord Africa (per allargarsi all'intero continente africano) una nuova ragione, che trova

Ma c'è un altro passaggio che ho citato prima, che è chiamato in causa in queste ore e di cui la vicenda dell'isola di Lampedusa diventa emblematico esempio. questo accordo, come dicevo prima, c'è quella di acquisire una collaborazione davvero positiva dello Stato libico nel contrastare questo fenomeno. Ad oggi gli esiti non sono soddisfacenti e certamente può essere invocato che si tratti di un accordo non ancora vigente in quanto non ancora ratificato; possiamo considerare la necessità di una fase di assestamento, perché questo accordo diventi impegnativo per le parti; ma ad oggi la politica del Governo che ha scelto questa collaborazione per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina non ha avuto il successo sperato. Abbiamo allora il paradosso di un accordo che sancisce riconoscimenti politici ma anche economici molto importanti e che non vede ad oggi restituito alcunché al nostro Paese in termini di sicurezza relativamente all'approdo degli immigrati clandestini, con l'isola di Lampedusa che diventa l'occasione anche di un confronto aspro nella comunità nazionale, sia per quanto riguarda le linee che devono ispirare la politica sull'immigrazione, tra il contrasto duro (ho letto oggi perfino "cattivo") e una linea anche di accoglienza intelligente che non determini incoraggiamento all'immigrazione clandestina. Ebbene, vi chiedo una cosa: che l'isola di Lampedusa non sia quella che paghi il prezzo per tutti. Comprendo che il Governo possa immaginare che una politica di contrasto debba evitare che da Lampedusa

di riservare un destino drammatico a quell'isola che si è costruita un futuro dignitoso in nome di un turismo che fa leva sulla salvaguardia ambientale e sulle capacità autoctone dei residenti.

che invece rimangono lì e rischiano di rimanerci per tempi insopportabili, devastando la convivenza civile di quella comunità e ovviamente anche le sue prospettive economiche. [**Presidenza della vice i princìpi di accoglienza umanitaria sempre, perché questo è in linea con la nostra Carta costituzionale; di garantire, se la politica è quella dei rimpatri immediati, che gli accordi bilaterali, a cominciare da quello con la Libia, siano efficaci e i rimpatri avvengano, come dice il Governo, nell'arco delle 24 ore e non dei 24 mesi; di garantire comunque a Lampedusa interventi risarcitori per il danno di immagine e quindi rilanciando il suo turismo, intervenendo in modo incisivo sui servizi primari, primi fra tutti scuola e sanità, intervenendo a sostegno dei suoi comparti economici, compreso quello della marineria, e garantendo all'isola, come segnale della comunità nazionale, collegamenti stabili che garantiscano intanto il diritto alla mobilità dei residenti. chiedo che il Governo sperimenti in modo veramente coerente su questo accordo la capacità politica nazionale e internazionale di sviluppare un'opera di cooperazione e di pace nel Mediterraneo che abbia come obiettivo lo sviluppo del fronte del Nord Africa, perché questa è l'unica condizione per disinnescare la miccia dell'immigrazione e per garantire pace e tranquillità in questo territorio. Per queste ragioni, che sono fondate molto sulla speranza, ma anche sulla buona volontà e sulla capacità del nostro Governo di attuare una politica estera in linea con gli interessi nazionali, quelli veri,

noi voteremo contro questa legge che autorizza la ratifica del Trattato italo-libico

Noi non siamo contrari a che l'Italia stipuli un accordo bilaterale con la Libia per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione clandestina, del traffico di migranti e di tutto ciò che attorno a questo traffico cresce in termini di finanziamento ad organizzazioni criminali criminali transnazionali che lucrano non meno di 24 milioni di euro l'anno solo sul traffico e sul trasporto dei migranti stessi. punto di vista, però, signora Presidente, c'è una differenza fra un trattato ed un accordo bilaterale.

un'intesa con il Governo tunisino finalizzata al rimpatrio dei 1.200 tunisini irregolari che sono presenti a Lampedusa.

poiché un Trattato, sotto il profilo giuridico-costituzionale, è la definizione di un sistema ordinamentale comune tra due Stati per la disciplina di alcune materie. due Stati d'intesa cedono una quota della propria sovranità nazionale, costruiscono insieme, perché hanno un interesse economico, geopolitico, culturale o di altro genere, un sistema giuridico conforme ai rispettivi ordinamenti costituzionali, ma un sistema giuridico comune che per quella determinata materia prescinde dall'applicazione della legislazione nazionale. Quindi, con la Libia abbiamo fatto un'operazione di questo tipo, che si giustifica se lo scopo del Trattato è quello di riparare i danni dell'esperienza coloniale italiana in Libia e se serve a chiudere quella pagina della storia del nostro Paese che, per la verità, non è stata tra le più felici. Se si vuole, però,utilizzare un Trattato per affrontare altre questioni altrettanto importanti, è necessario che il contenuto dello stesso sia coerente con lo scopo che si vuole perseguire. Noi in questo caso stiamo facendo un pasticcio,

e discipliniamo, in una sorta di zibaldone, tanti aspetti in cui alla fine ciò che emerge è la totale cessione della sovranità nazionale del nostro Paese su alcune questioni pagate dai contribuenti italiani con l'addizionale sulla tassa del gas che colpirà solo l'ENI (perché l'articolo che prevede le coperture ha una sigla ben precisa) e quindi tutto ciò sarà scaricato sul consumatore finale, quindi sui cittadini italiani. Per fare un'opera di pattugliamento congiunto alle frontiere libiche, cioè di personale di forze militari o di polizia italiane insieme a quelle libiche (queste ultime pagate dall'Unione europea, le nostre pagate dai cittadini italiani con una tassa *ad hoc*), per fare questa operazione (ora vedremo la complessità e la praticabilità della stessa), diciamo che i passi avanti che la trattativa che l'Italia ha fatto (e va rivendicata a merito dei tanto vituperati Governi della prima Repubblica e non solo), i passi avanti che sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, dell'accettazione della Convenzione di Ginevra e delle convenzioni internazionali e dell'integrazione del rapporto bilaterale fra l'Unione europea e la Libia (questo è il successo politico e internazionale dell'Italia), i passi in avanti che sono stati fatti si fermano ad un certo punto; si fermano al punto in cui si cristallizza nel Trattato

anzi può continuare a fare ciò che fa in Libia, e tutto questo con l'accordo italiano. L'accordo italiano si traduce nella circostanza che non riusciamo a comprendere quali siano o quali saranno le regole d'ingaggio che le forze italiane che saranno chiamate a pattugliare le frontiere libiche dovranno applicare, ossia se sono le regole del diritto interno interno italiano, se sono le regole del diritto internazionale o se sono le regole del diritto libico. Immagino che non siano le regole del diritto libico, altrimenti credo che avremo difficoltà anche a reclutare il personale. Ma non solo: si fa un'operazione che, sotto questo profilo e per quanto riguarda il contrasto all'immigrazione clandestina, è inutile, se non pericolosa. facendo quattro conti, il pattugliamento delle frontiere libiche e il respingimento alla frontiera libica- perché di questo si tratta - deve essere fatto - io immagino - secondo le regole previste dal diritto internazionale e dal diritto italiano;

stanno le cose, è evidente che la prima cosa che le forze italiane dovranno fare, considerato che molta di questa gente viene da lunghe traversate nel deserto, è prestare assistenza - così come avveniva

rotte; e poiché non credo che abbiamo intenzione di presidiare o pattugliare (salvo che non abbiamo in testa una seconda esperienza coloniale) tutti i confini dei Paesi interessati, faremo spendere ai cittadini delle risorse in maniera inutile.

per consentire a quello Stato di applicare regole ed esercitare funzioni e competenze proprie di uno Stato moderno e di diritto anche nel contrasto all'immigrazione clandestina, un altro conto è sostituirsi a quelle forze di polizia.

con l'Unione europea sulla materia. Da ultimo, signora Presidente, facciamo un Trattato con cui poniamo fine ai danni del colonialismo e diamo le briciole ai nostri connazionali che sono stati espulsi e i cui beni sono stati confiscati. Non c'è una parola sui beni degli italiani espulsi

se non a fare un po' di propaganda ai fini del contrasto all'immigrazione clandestina. Se mi è consentito sottolinearlo, sarà anche "opaco", perché, nel momento in cui non si stabiliscono le regole con cui si scelgono le imprese alle quali si danno 200 milioni di euro l'anno per realizzare opere in Libia (alla faccia della libera concorrenza!), si fa un danno anche all'economia e alle imprese italiane che non concorrono liberamente per l'aggiudicazione di queste gare.

La discussione ha permesso di mettere in luce le tante ombre che l'accordo presenta. Voglio precisare che la posizione espressa non è strumentale o meramente ostruzionistica nei confronti dell'operato del Governo. Anche nell'altro ramo del Parlamento, infatti, il Gruppo Italia dei Valori si è attestato sulla linea del confronto sul merito del provvedimento, avendo ben presenti le ragioni che hanno spinto gli ultimi Governi, e non solo quello attuale, a trattare un accordo con la Libia. Vorrei premettere, inoltre, che l'Italia dei Valori ritiene auspicabile, anzi fondamentale, per l'Italia lo sviluppo di una rete di relazioni bilaterali e di un sistema di accordi multilaterali nell'area del Mediterraneo. Il Mediterraneo rappresenta una risorsa imprescindibile per tutti, sotto l'aspetto culturale, economico e sociale, e l'Italia, per la sua posizione geografica e per le relazioni pregresse coltivate dai Governi che si sono succeduti, rappresenta un attore fondamentale e privilegiato, anche nel consesso degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di sviluppare una politica di crescita democratica dell'area. Nei rapporti specifici con la Libia, il nostro Paese ha gli strumenti per potere instaurare una sempre più proficua politica di vicinato, e l'impegno in tale senso è innegabilmente motivato anche dalle obbligazioni che derivano dall'eredità del passato coloniale. Pertanto, arrivare ad un accordo con la Libia è senza dubbio un passo importantissimo, non soltanto per chiudere un capitolo della storia, ma anche per avviare un processo che avvicini all'area democratica e pacifica dell'Europa anche Governi, come quello libico, sulla cui legittimità democratica il nostro Gruppo - e l'opinione internazionale - nutre forti dubbi. Questa logica di influenza positiva, di *moral suasion*, così dire, che l'Italia avrebbe dovuto esercitare nei confronti della Libia per spingerla verso un processo democratico quando ha negoziato il Trattato in oggetto non è è un'idea peregrina dell'Italia dei Valori, ma è la logica sottostante a tutta la politica di allargamento dell'Unione europea. Infatti, nei Protocolli di adesione per i Paesi che intendono entrare nella Comunità, c'è l'obbligo di condividere l'*acquis communautaire* dell'Unione, ossia quei principi di stato di diritto, di giustizia, di politica economica su cui si basa tutto il progetto europeo dal 1957. Non è dunque sull'opportunità di concludere un Trattato di amicizia con il Governo della Libia che esprimiamo la nostra contrarietà, ma sul contenuto di questo Trattato e soprattutto sulle modalità con le quali il Governo in carica ha condotto i negoziati e raggiunto un accordo! Infatti, come dicevo all'inizio, l'Italia dei Valori concorda su atti bilaterali e multilaterali che portino in sé anche aspetti di evoluzione democratica, per molti aspetti questo accordo è unilaterale. Lo è nel dare finanziamenti per 5 miliardi in opere infrastrutturali alla Libia che verranno sviluppate da imprese italiane selezionate non si sa su quale base; base; è unilaterale nello strutturare un sistema di controllo delle frontiere interne del Paese firmatario, che sarà basato su risorse italiane ma anche europee, senza che, per queste ultime, sia stato dato un preciso ed ufficiale avallo da parte della Commissione europea; è unilaterale nello stabilire la somma da destinare come indennizzo nei confronti di cittadini italiani, enti e società che nel 1970 si sono ritrovate senza una lira, senza dignità, senza nulla; è unilaterale perché rispetto alle ampie concessioni che il Governo ha fatto alla Libia niente è stato ottenuto in cambio. Certo, non è stato ottenuto l'obbligo del rispetto dei diritti umani dei migranti. Proprio per questo hanno

questi atti sono commessi da Paese in guerra o dittatoriali come Etiopia, Sudan, Eritrea, Somalia; non è garantito alcun diritto. Per questo alla Libia non può essere affidato con tanta noncuranza e superficialità il compito di fermare i migranti.

premio Nobel Dario Fo, cioè una commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulle modalità di controllo dei flussi migratori in Libia. Questa è la richiesta che centinaia di intellettuali hanno firmato. di alcuni emendamenti, la volontà di istituire una commissione, che non comporti alcun onere a carico dello Stato, preposta al controllo e al monitoraggio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che non dovrebbero mai essere compromessi per motivi di opportunità politica o interessi economici. - vi chiedo, colleghi - mantenere costante vigilanza sul rispetto dei diritti umani da parte di un Paese che non ha nel proprio ordinamento la possibilità di richiedere il diritto d'asilo, che non ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti dei rifugiati, che è oggetto di numerose denunce per violazioni da parte di Amnesty International? Definisco poi questo Trattato unilaterale sulla base di riflessioni relative a ciò che sancisce il diritto internazionale. La già sottolineata incompatibilità tra quanto previsto all'articolo 4, comma 2, di questo trattato e il dettato dell'articolo 5 del Trattato NATO, vale a dire che si promette di non esercitare alcun atto ostile contro la Libia, ma più rilevantemente ci si impegna a non concedere l'uso delle basi militari presenti sul nostro territorio per qualsiasi atto ostile contro la Libia, si basa infatti su ciò che il diritto internazionale sancisce, non su fobie o su fobie o voli pindarici dell'Italia dei Valori. So bene che a tal riguardo il Governo, nella persona del Ministro degli affari esteri, ha più volte rappresentato la prevalenza del dettato del Trattato NATO e la sua non modificabilità alla luce di questo accordo bilaterale. Di queste precisazioni l'Italia dei Valori si rallegra, ma converrete con me che, se tutti gli Stati che aderiscono alla NATO regolassero i propri rapporti diplomatici con altri Paesi con testi di questo tenore, il risultato non sarebbe poi così glorioso come il Governo e la sua maggioranza vorrebbero rappresentare. Infatti, la prevalenza del Trattato NATO che vi ostinate a sostenere non si basa su veridicità giuridica, poiché poiché - ma non dovrei insegnarvelo io - il richiamo fatto nel Trattato al «rispetto dei principi della legalità internazionale» nulla può contro il meccanismo base del diritto internazionale per cui ogni atto pattizio, come il Patto atlantico, perde di efficacia al subentrare di un successivo atto pattizio come quello firmato con la Libia. forza per la difesa della sicurezza internazionale non rientra in nessuno dei principi dello *ius cogens* che sono sovraordinati al diritto convenzionale. *Ergo*, nel caso in cui una operazione multilaterale dovesse essere attivata nei confronti della Libia a seguito di un attacco della stessa ad un Paese NATO, l'Italia potrebbe trovarsi nella situazione imbarazzante di non poter cooperare all'azione multilaterale in quanto vincolata dal Trattato che oggi ci impegniamo a ratificare. Vorrei riprendere la generosità di concedere 5 miliardi di investimenti per giustificare la quale il presidente Berlusconi ha propagandato i vantaggi di ricevere gas, petrolio dalla Libia e di fermare l'immigrazione clandestina. Ma per far credere che questo accordo risolva l'emergenza migratoria verso le nostre coste, che spero voti come noi), è una truffa. Gli sbarchi di immigrati che partono dalla Libia sono gestiti da mercanti di schiavi che trovano la complicità di settori collusi della polizia libica e i numeri degli ultimi mesi smentiscono meglio di tutti questa illusione, dato che il numero di clandestini giunti sulle nostre coste ha toccato il record proprio nei mesi successivi all'accordo del 30 agosto. Concludo quindi, signora Presidente, pur riconoscendo le necessità di dover trattare con un Paese dalla risaputa e storica inaffidabilità, il Gruppo Italia dei Valori, come ha ben sostenuto anche alla Camera il presidente Di Pietro, non può non esprimere parere contrario circa un metodo di gestire i rapporti diplomatici e la politica estera in generale al quale, purtroppo, questo Governo ci sta abituando (già con la crisi georgiana), dimostrando di considerare la politica estera strumento di rapporti personali, e non diplomatici, tra i *leader* degli Stati al posto dei loro Governi. E concludo: questa considerazione, vorrei sottolinearlo, si inscrive nella linea che anche il nostro capo dello Stato, il presidente Napolitano, ha più volte dettato, a partire dalla crisi georgiana, quando, in un comunicato ufficiale dalla Finlandia, ha ribadito che la politica estera la fanno gli Stati, gli Stati e solo gli Stati! L'amicizia personale non c'entra nulla, altrimenti si svilisce il senso dello Stato. Non mi resta altro da dire, signora Presidente, onorevoli colleghi, se non, con una certa amara ironia, che, a seguito della ratifica di questo accordo, i giornali potrebbero titolare le prime pagine di domani mattina, richiamando il nostro inno nazionale e mutandone soltanto il soggetto, "La Libia s'è desta!". Ma l'Italia? L'Italia si è al contrario piegata ad una falsa *realpolitik*? Lascio a voi la risposta, colleghi e Governo. Il Gruppo Italia dei Valori ha già la sua risposta e per questo vota no, vota no con forza, vota no convinta alla ratifica di questo Trattato.

Signora Presidente, noi non siamo molto abituati a letture capziose o arzigogolate. Guardiamo un po' più in faccia la realtà dei fatti. Dobbiamo dire una cosa, cari colleghi: forse, per la prima volta dopo tanti anni, si parla un'altra lingua. Dopo anni di tensione con la Libia, possiamo leggere il titolo del Trattato dove si parla di amicizia e di cooperazione. Potremmo dire che l'oggetto sostanziale di questo Trattato è un recupero dei rapporti con la Libia; caratterizzati da continue crisi, fin dal 1969, da quando si insedia al potere Muammar al Gheddafi**.** Infatti, l'anno successivo gli italiani vengono cacciati dalla Libia, le proprietà italiane vengono confiscate,

La risposta della Libia è la seguente: siccome l'Occidente è accomunato bisogna mandare un segnale all'Europa. Qual è il posto più vicino? L'Italia. Forse è soltanto per una questione balistica che il missile indirizzato a Lampedusa non esplode e non produce, Il Senato ne avrebbe potuto avere un grande danno: forse oggi non sarebbe presente l'unica parlamentare che mai abbia espresso l'isola, la senatrice Maraventano, che ci sembra del resto molto impegnata sul fronte che poi il Trattato oggettivamente affronta.

la comunità internazionale la obbliga a consegnare almeno i presunti responsabili. Quando è che cambiano questi rapporti? La normalizzazione avviene, più o meno, nel 2003, quando la Libia finalmente un accordo con la comunità internazionale e firma al Consiglio di sicurezza dell'ONU un atto con il quale si impegna a non partecipare più a nessun atto di terrorismo ed a rinunciare per sempre a programmi di costruzione di armi di distruzione di massa; inoltre, essa si impegna a concedere un risarcimento dei danni a tutte le vittime degli attentati che l'hanno vista più o meno coinvolta.

Da quel momento anche i rapporti con l'Italia divengono più distesi; infatti, si stringono accordi bilaterali sul turismo, sulla cooperazione culturale, sulla protezione degli investimenti dei reciproci Paesi. Sono però tutti pezzetti, è una specie di mosaico, che solo oggi va a creare un quadro di una certa compiutezza con l'accordo attuale. Cosa potremmo dire noi,

Ci costa qualcosa? Ahimè, tutto ha un prezzo. Il costo dell'operazione, sulla carta, sembra importante: 5 miliardi di dollari.

Verranno gestiti dall'Italia selezionando imprese esecutrici dei lavori che opereranno in Libia, per un ammontare di investimenti pari, nel ventennio, a 5 miliardi di dollari. È molto diverso fare un'iniezione keynesiana interventista, sul territorio o fuori del territorio, quando sono sempre soggetti italiani a partecipare, creando reddito e pagando le imposte nel nostro Paese.

Le depredazioni non sono cose buone. Metà dei musei europei è piena di materiali più o meno prelevati; il restituire manoscritti o reperti archeologici dichiaratamente di proprietà dello Stato libico ci sembra quasi un gesto di dovuta generosità Una cosa importante che nessuno ha avuto il coraggio di sottolineare è che c'è una contropartita:

l'incasso del mancato introito e guadagno, che si può stimare in 250 milioni di euro, che rientreranno immediatamente in Italia, nelle casse di imprese Scusate se è poco il fatto che la Libia si dichiari non ostile nei confronti dello Stato italiano e che non si possano usare i reciproci territori per attività ostili all'altra parte.

che riguarda il rafforzamento della collaborazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e l'immigrazione clandestina.

soprattutto quelle terrestri - verranno gestite e controllate da forze militari italiane, saremo ancor più sicuri che esse verranno gestite in modo attento, a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini italiani. se a voi sembra poca cosa il fatto che la Libia firmi un trattato in cui si impegna a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo e dunque, sostanzialmente, gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani:

non si era mai vista un'operazione così importante costare così poco alla comunità. Nessun cittadino pagherà un solo centesimo di euro per questa operazione. Se andiamo a leggere la parte che riguarda la copertura finanziaria, tratta di una specie di Robin Hood *tax* perché pagheranno i costi di questa operazione soltanto quelle imprese e società commerciali, residenti in Italia, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi e che hanno e che hanno una capitalizzazione superiore ai 20 miliardi di euro. Signori, forse sbaglieremo, ma a conti fatti soltanto l'ENI rientra, per cui tutti i cittadini ne beneficeranno e soltanto un'impresa, con un'addizionale del 4 per cento, si sobbarcherà i costi.

15 anni che ha interessato diversi Governi di questo Paese, una vicenda che è stata accompagnata da una progressiva normalizzazione dei rapporti bilaterali e che si è via via nutrita dell'intensificarsi dei rapporti economici, tra questi due Paesi, come si evince anche dalle notizie di alcuni importanti investimenti che sono intervenuti anche di recente nel nostro Paese. Come è stato qui ricordato nel corso della discussione, tutto ha inizio quando le Nazioni Unite decidono di porre fine al regime sanzionatorio a seguito della decisione dello Stato libico di accettare l'autorità internazionale sul caso Lockerbie. Accadde allora, e vorrei che venisse ricordato in questa circostanza, che l'Italia fu il primo Paese occidentale ad interrompere l'embargo e ad avviare quelle procedure che oggi si concludono, con una intesa preventiva con l'allora Governo degli Stati Uniti. Dico questo perché quella scelta avveniva nel solco di una scelta di politica estera che assume, e noi riteniamo che debba continuare ad assumere, il tema della stabilità e della sicurezza del Mediterraneo come scelta strategica, accanto alla scelta di dare nuovo vigore a quel rapporto euro-africano sul quale io credo che l'Europa debba puntare molto nel futuro. Tutti gli interventi del nostro Gruppo, così densi di argomenti, partivano comunque da un dato fondamentale: la Libia evoca una delle pagine più ingloriose del colonialismo italiano, un'esperienza coloniale che si è accompagnata anche a crimini contro la popolazione civile, crimini che hanno lasciato segni indelebili e anche chi oggi sta ricostruendo quella vicenda storica, il tanto tempo trascorso, resta davvero ancora segnato da quei crimini. Riconoscere queste responsabilità, risarcire quel Paese per queste responsabilità, io credo che sia un atto che fa onore al nostro Paese. Non è un caso che tanti altri Paesi, vittime del dominio coloniale, stiano prendendo ad esempio la nostra esperienza per avviare anche loro iniziative di questo tipo.

nel favorire una ripresa dei rapporti tra la Libia e gli Stati Uniti, che sono diventati importanti, soprattutto su questioni che attengono alla sicurezza e alla lotta al fondamentalismo islamico: è un merito del nostro Paese. Con questo Trattato, dunque, si consolida un partenariato economico che ha rappresentato e rappresenta una risorsa importante per il nostro Paese. Non si può trascurare

e nei nostri interventi e negli ordini del giorno che abbiamo presentato lo abbiamo ribadito. Penso ai temi della quantificazione finanziaria

A tale proposito, il senatore Livi Bacci ha detto cose estremamente importanti in questa discussione: non bisogna farsi nessuna illusione sugli effetti di questo accordo sul contrasto all'immigrazione clandestina, tanto più in presenza di un fenomeno che sta assumendo dimensioni davvero consistenti, che presenta aspetti terribilmente drammatici e pone anche a noi l'esigenza di un approccio che non può essere quello che risuonava nelle parole ieri pronunciate dal Ministro dell'interno di questo Paese, che ci hanno lasciati interdetti e anche indignati. senza ipocrisie e infingimenti: una politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina non la si effettua nel Mediterraneo. I Paesi che si affacciano sulla riva meridionale di questo nostro mare sono di transito dell'immigrazione e allora o si porta avanti questa politica insieme ad essi, in un rapporto proficuo con quelli africani, oppure questa sarà priva di qualsiasi risultato. Per intenderci, né le politiche di contrasto né quelle di più forti controlli del fenomeno daranno risultati se non saranno accompagnate da accordi di riammissione con i Paesi di

Tra l'altro, la totale mancanza di fondi per la cooperazione nella legge finanziaria, tanto più in coincidenza con la Presidenza del G8 che spetterà al nostro Paese, rischia di produrre tanti begli annunci, magari anche di carattere telefonico, e pochi concreti risultati. In questa visione, abbiamo collocato le questioni poste nell'ordine del giorno proposto dal nostro Gruppo abbiamo voluto e intendiamo in questa sede, ancora una volta, richiamare il Governo a pretendere - in virtù delle intese bilaterali, contenute nell'articolo 19 del Trattato - la garanzia del rispetto dei diritti umani nei confronti dei migranti e delle norme di diritto internazionale circa la protezione dei rifugiati. Dunque, noi voteremo a favore di questo Trattato. Un rinvio - vedete oggi suonerebbe come un incomprensibile atto di ostilità nei confronti di quel Paese. Si può consolidare un quadro di relazioni, non solo di partenariato energetico, ma anche per le nuove opportunità di mercato che si aprono per il nostro Paese e pure sul piano culturale. Non vorrei che si dimenticasse che la Libia è l'unico Paese arabo in cui si parla italiano. Un riscatto storico, dunque, una utile e lungimirante operazione diplomatica verso il mondo arabo. Un Trattato che corrisponde agli interessi generali dell'Italia e che dunque, con questa impostazione, noi sosterremo con il nostro voto. Signora Presidente, colleghi, c'è un accenno che è emerso poco nel nostro dibattito di questo pomeriggio vale a dire la valenza che questo Trattato di amicizia tra la Libia e l'Italia ha non non soltanto nell'ambito delle relazioni internazionali tra i due Paesi che hanno firmato il Trattato, ma anche nei rapporti con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e nel contesto africano: questo è un Trattato destinato probabilmente a lasciare dei segni anche nei Paesi che sono vicini ma non fanno parte del Trattato stesso. Credo che questo Trattato costituisca il punto di arrivo di negoziazioni portate avanti da Governi di diverso colore politico e già questo è un segno di una continuità di intenti dell'impostazione della politica italiana rispetto alla Libia negli ultimi venti anni. Il fatto che più Governi si siano succeduti, di colore politico diverso, ma abbiano tutti sottolineato la necessità di procedere a questo Trattato, con punti di vista diversi, con anche risultati diversi, con un dibattito diverso, che ha per esempio portato portato l'onorevole D'Alema a dire che questo è un Trattato che si doveva fare perché è utile anche all'Italia. Questo che è stato suggellato dal Governo in carica è comunque un fatto politico importante. L'omogeneità della visuale nel variare delle maggioranze politiche deriva evidentemente dalla condivisione delle opportunità per il nostro Paese di voltare pagina rispetto al passato coloniale e di procedere in un'ottica di leale collaborazione con un Paese, quale la Libia, vicino geograficamente e legato storicamente a noi. Del resto, ogni Trattato internazionale non può che disciplinare un assetto di interessi frutto di sedimentazione passata, indicando un intento programmatico per il futuro. dicevo pure in Commissione, la caratteristica di un Trattato è anche di costituire il punto di partenza di un lavoro, di una mediazione a risultati e a condizioni migliori rispetto a quelli di partenza. Il Trattato costituisce un significativo passo in avanti nei rapporti tra Italia e Libia, per esempio, con il passaggio dal comunicato congiunto italo-libico del 4 luglio 1998 ad un vero e proprio accordo di amicizia, partenariato e collaborazione.

Al di là, poi, del rilevante valore simbolico del Trattato di amicizia, occorre peraltro sottolineare che nei contenuti le protratte trattative con la Libia hanno condotto ad un accordo che equilibra le esigenze principali dei due Paesi: da un lato, infatti, si tiene conto che la Libia per noi è uno dei principali partner commerciali soprattutto nella politica energetica; dall'altro, le opere infrastrutturali di cui necessita la Libia saranno costruite da imprese italiane, fatto che costituisce la premessa per rafforzare le già intense relazioni industriali. E questo progresso nelle nostre relazioni internazionali è un altro passo che non ho sentito evocato nel nostro dibattito. Tra le problematiche affrontate dal disegno di legge in esame di maggiore delicatezza segnalo la definizione del contenzioso relativo agli indennizzi per gli espropri subiti da cittadini e imprese italiane da parte delle autorità libiche, quale capitolo che completa la soluzione delle questioni ancora aperte e connesse al periodo coloniale e delle correlative posizioni dei due Stati. Sono d'accordo con le osservazioni fatte anche dall'opposizione sulla necessità che questo capitolo venga chiuso nel più breve tempo possibile. Un ulteriore ambito in cui la cooperazione tra Italia e Libia sarà imprescindibile è quello del contrasto all'immigrazione irregolare in seno al bacino del Mediterraneo. E' infatti quanto mai necessaria una coordinazione degli interventi tra Paesi di provenienza dei flussi migratori, aree geografiche di transito e Paesi di destinazione intermedia e finale dei migranti. Vorrei conclusivamente fare un'annotazione di ordine generale sul fatto che il Trattato di amicizia, così come strutturato, definisce le premesse per un punto di partenza delle principali problematiche su cui la collaborazione italo-libica si svilupperà, rinviando tuttavia ad ulteriori accordi, scambi di lettere e comitati la concreta definizione e attuazione delle pattuizioni. Nel dichiarare il convinto sostegno del Popolo della Libertà al Trattato in esame, formulo quindi l'auspicio che il positivo clima che ha consentito la sottoscrizione dell'Accordo persista anche nelle successive fasi di attuazione e specificazione dei patti, e che la collaborazione tra Italia e Libia prosegua su binari nuovi nel senso di un rinnovato spirito di amicizia che si basa sul superamento delle esperienze storiche trascorse. *(Applausi Presidente, colleghi, vi chiedo un supplemento di pazienza ed anche di immaginazione. Immaginate di essere un libero pensatore, una donna, un cristiano, un ebreo e di trovarvi in Libia. Immaginate un Governo che ritiene di dover dare dei soldi a quello che non vi fa essere quello che voi volete essere e lo

premete il tasto verde a favore di questo Trattato. Gheddafi non ha mai mantenuto una sola volta la parola data nei confronti dei suoi *partners* internazionali e voi non soltanto gli date dei quattrini, ma glieli date per sopprimere la libertà, i diritti umani e lo Stato di diritto in quel Paese.

è un altro Trattato e in particolar modo lo ricordo ai colleghi del centrosinistra. È un altro Trattato, ma purtroppo l'interlocutore è lo stesso, è Gheddafi, quello che non rispetta i diritti umani, quello che permette la tortura, la pena di morte, la violenza sulle donne e anche sui bambini, quello che viola i diritti dei rifugiati. Già, perché la Libia è uno di quei pochi Paesi che non hanno sottoscritto e firmato la Convenzione relativa

Dichiaro aperta la votazione.